Signora Presidente, ci tengo a intervenire perché voglio sottolineare che stiamo parlando di un tema assolutamente importante quale quello della sottrazione internazionale dei minori e di come il nostro Stato su questo stia

che essa venga rafforzata anche nella sua funzione di relazione tempestiva e costante con le famiglie coinvolte. Al fine di facilitare la relazione tra la *task* *force* e le famiglie, prevediamo che un membro del Governo

delle sentenze e il sostegno dell'attività alle frontiere per evitare l'uscita dei bambini sottratti nasce dal fatto che non c'è uno specifico reato per quanto riguarda la sottrazione internazionale dei minori. Individuiamo, quindi, senza automatismo, la preclusione dell'applicazione delle circostanze generiche

in favore di un'iniziativa di coordinamento tra le legislazioni nazionali in materia di diritto di famiglia e a continuare a favorire in ambito comunitario ogni iniziativa utile a migliorare la comunicazione tra il mediatore europeo e le Autorità centrali degli Stati membri;

L'ultima questione - ma non ultima per importanza - riguarda la necessità di favorire, quanto alla normativa sovranazionale (su cui stiamo lavorando, in modo particolare nella fase di revisione del Regolamento di Bruxelles II), una rivisitazione all'attuale formulazione dell'articolo 13, che spesso viene utilizzato

che ha portato alla predisposizione di un testo unitario sul tema dei minori sottratti. È un tema importante sul quale il Governo, alla luce di questa richiesta unanime del Senato, intende impegnarsi, ragion

bambini, impegna il Governo ad avviare, nel quadro delle ulteriori iniziative già intraprese, un'attività di monitoraggio volta a contrastare, sul territorio italiano, lo sfruttamento di minori da parte delle organizzazioni criminali.

signora Presidente, anche perché questa mattina ci siamo incontrati con tutti gli altri proponenti e rispetto a questa mozione, che porta alla ribalta la questione di minori di cui non si ha più notizia (si parla di oltre 5.000 solo in Italia e 26.000 in tutta Europa), abbiamo abbiamo concordato un testo in cui si impegna il Governo a monitorare il fenomeno, e quindi, per quanto possibile, ad affrontarlo. È un tema di particolare importanza e urgenza, un dramma nel dramma; quindi, ringrazio sia

Ho già presentato un nuovo testo sottoscritto anche dai colleghi. finestra"). Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Marie Curie» di Napoli. Benvenute e benvenuti al Senato. Grazie Presidente,

È un fenomeno, questo, che a sentirne parlare così sembra qualcosa di sporadico. In realtà i casi sono numerosissimi e probabilmente non si riesce nemmeno ad averne contezza. È un fenomeno, tra l'altro, crescente dovuto all'incremento dei flussi migratori perché molto spesso, colleghi, la sottrazione del minore avviene proprio in sede di rottura di rapporti di tipo affettivo

Tra l'altro, la difficoltà si presenta anche perché in molti Paesi dove viene portato il minore vi è anche la possibilità, in base alla legislazione nazionale, di poter portare con sé il proprio figlio, magari aiutati da una normativa diversa da quella italiana che consente di avere una tutela.

che nella normativa, sia a livello nazionale che internazionale, viene sottolineato il superiore interesse del minore e non si sta parlando soltanto di una dizione squisitamente giuridica perché «superiore interesse del minore» significa che nel momento in cui vi è un conflitto fra genitori che si sono separati, si sono lasciati, e dove ognuno, ovviamente, ascrive a sé il diritto di portare con sé il figlio, di curarlo e farlo crescere nel proprio modo nel proprio Paese, ricordare che sicuramente quello che deve essere valutato è solo il benessere del bambino. Questo fondamentale principio è stato più volte ricordato nella normativa internazionale

si auspica e si chiede che non resti solo una dichiarazione d'intenti, e che si esplichi nella pratica in provvedimenti effettivi.

la possibilità di bloccare il rimpatrio del minore ogni qualvolta vi siano delle situazioni definite intollerabili o pericolose.

Ma la grande difficoltà è che la sanzione penale ivi prevista, ossia un massimo di quattro anni della pena edittale, comporta l'inapplicabilità di istituti fondamentali in fase istruttoria delle indagini. Infatti non sarebbero ammesse né intercettazioni telefoniche ambientali né l'applicazione della custodia cautelare.

che gestisca una forma di cooperazione tra tutte le istituzioni che vengono coinvolte in queste complesse procedure, con aspetti burocratici, tra l'altro, molto difficili.

La figura di riferimento della *task force* italiana sarà anche chiamata a coordinarsi con questo mediatore europeo e sarà un ulteriore rafforzamento dell'aiuto nel percorso. Devo dire che approvo con molto favore anche quanto detto al punto 10), con riferimento alla riformulazione dell'articolo 13, perché vedo che spesso molte Nazioni straniere fanno difficoltà

non sempre quest'Assemblea scrive delle belle pagine di politica e soprattutto non sempre si registra una così ampia e sentita condivisione. Oggi noi scriviamo una bella pagina della politica. Oggi noi diamo a quelle persone e a quelle famiglie, che non sanno più dove è il loro figlio o la loro figlia, un senso di grande protezione. Lo Stato oggi dice a queste famiglie: io sono al vostro fianco, io vi proteggo, io farò il percorso insieme a voi. Fino ad oggi, in maniera anche estremamente professionale, i Ministeri si sono avvalsi delle loro competenze e delle loro responsabilità per far pressione rispetto ad altri Paesi che trattenevano in modo illecito i bambini italiani.

facciamo un passo ulteriore: il passo di un Governo responsabile, di uno Stato responsabile, che mette a disposizione un punto di riferimento che farà da coordinamento. la buona volontà cammina sulle gambe di persone responsabili; ma insieme si può fare molto di più. che chiediamo ai tre Ministeri competenti, il Ministero della giustizia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno, affinché insieme possano trovare soluzioni e spingere maggiormente per riavere a casa i propri figli.

linee guida per le procure, le prime ad accogliere il disperato appello di genitori disperati; linee guida per le nostre ambasciate, affinché anche loro, che rappresentano l'Italia, possano essere dei soldati attenti e possano fare le giuste pressioni, laddove è possibile, per riportare a casa questi bambini. Parlamento, pertanto, oggi scrive una bella pagina e diventerà anche motivo di orgoglio ogni anno vedere come questo nuovo e rinnovato impegno del Parlamento porterà i suoi frutti;

Lei oggi in quest'Assemblea scrive insieme a noi questa bella pagina e tanti genitori le saranno grati di ciò, perché lei oggi rappresenta lo Stato e dà un parere favorevole a questa nuova azione. È un ben cominciare per lei occuparsi di minori, di bambini scomparsi e sottratti illecitamente, bambini ai quali oggi diamo una speranza di ritorno a casa.

Presidente, colleghi, il rapporto genitori-figli è un legame prezioso, speciale, che andrebbe preservato e tutelato in qualunque situazione. Se ne è parlato molto durante l'approvazione del disegno di legge sulle unioni civili quando, attraverso il tentativo da parte del Governo e della maggioranza (tentativo peraltro miseramente fallito) d'introdurre nel nostro ordinamento l'istituto della *stepchild adoption* anche per le coppie omosessuali, si è più volte fatto strumentalmente

e che in quest'Aula oggi sottoscriviamo ancor più con l'approvazione della mozione all'ordine del giorno. Il tema che abbiamo finalmente iniziato ad affrontare da giovedì scorso è sicuramente spinoso, perché il dolore vissuto da tutti quei genitori che si vedono sottratti inaspettatamente i propri figli dal coniuge o congiunto non può essere ignorato e richiede un impegno massimo e quanto più possibile condiviso da parte delle forze politiche presenti in quest'Aula. È in questa direzione che abbiamo lavorato da questa mattina per arrivare a una mozione il più possibile condivisa. L'obiettivo della nostra discussione e della mozione che ci apprestiamo ad approvare deve essere solo uno: la tutela ovvero il rapido ripristino del legame genitore-figlio. Le sofferenze che hanno patito genitori che subiscono la sottrazione internazionale dei propri figli da parte del coniuge e i costi che essi sostengono per le conseguenti operazioni di ricerca sono indicibili e non quantificabili. I genitori vittime di questi drammi agiscono quasi sempre da soli e non possono contare su un riferimento istituzionale certo ed efficiente, quindi subiscono la frammentarietà dell'azione dei vari organismi istituzionali competenti in materia, che limitano di fatto l'efficacia dell'attività investigativa di gran parte delle procure e polizie giudiziarie presenti sul territorio nazionale, con pochissime eccezioni come quella della Provincia di Vicenza.

all'interno del Governo, con un membro del Governo che si faccia carico di questo coordinamento e che relazioni annualmente al Parlamento, ci sembra essere una decisione davvero di buon senso e doverosa verso la sofferenza di queste famiglie. Le criticità maggiori sono infatti rappresentate dalla difficoltà, molto spesso insormontabili, che i genitori coinvolti in queste tragiche vicende riscontrano quotidianamente nel comunicare con le istituzioni,

Questo punto, specificamente chiesto da noi del Movimento 5 Stelle, è ritenuto importantissimo, perché le famiglie non possono restare in un limbo e in un'assoluta inconsapevolezza di quanto si sta portando avanti e di cosa sta sta accadendo, anche qualora la *task force* si adoperi per il ritrovamento del minore. È giusto che le famiglie siano costantemente informate ed è importante che

per la soluzione del caso e sulle difficoltà riscontrate che rallentano la positiva chiusura del caso con il ritorno del minore nel Paese d'origine. Avere informazioni è sempre e comunque un diritto ed è sempre qualcosa di importante per un genitore che vive nell'ansia di poter riabbracciare il proprio figlio, del quale ha avuto cura cura dalla nascita fino al giorno della sottrazione. Allo stesso modo appare ineludibile procedere al rafforzamento del quadro sanzionatorio, iniziando a considerare come necessario l'inserimento della fattispecie di sequestro del minore nell'ambito dei delitti contro la persona e la libertà personale, nonché l'innalzamento delle pene edittali che, essendo attualmente di quattro anni, risultano insufficienti per la messa in atto ed efficacia di alcuni strumenti di prova come le intercettazioni ambientali e telefoniche, elementi indispensabili per individuare il minore sottratto e riportarlo il più rapidamente possibile nel proprio Paese d'origine. Su questo ci adopereremo, e siamo fiduciosi che ci sarà, a breve, una una trattazione dei disegni di legge che chiedono all'unanimità, anche in questo caso, come è stato fatto per la mozione, la modifica della legislazione. Altresì indifferibile, e pertanto condivisibile, nell'ottica del necessario superamento della frammentarietà, è il dialogo nell'azione degli organismi operativi per assicurare ai diversi soggetti istituzionali competenti in materia un reale coordinamento, sia nell'ottica della prevenzione del fenomeno che nell'ottica dell'orientamento e del sostegno alle persone coinvolte, nell'interesse primario dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero. Per quanto riguarda l'impegno 8), auspichiamo che l'attività di controllo alle frontiere si intenda come una tempestiva risposta alla presentazione di denunce o segnalazioni e non una restrizione della libertà di circolazione, perché questa mozione resti finalizzata alla tutela dei minori e non ad altri scopi, che spesso abbiamo visti inseriti in ottimi provvedimenti che solo all'apparenza sembravano tali.

Stavo dicendo che oggi è una giornata importante per le famiglie, per i genitori e per i bambini sottratti a livello internazionale. Quando il Parlamento vuole, a prescindere dalle bandiere e dai paletti politici,

Il problema della sottrazione internazionale dei minori risale a tempi antichi, tant'è che la Convenzione dell'ONU del 1980 e la Convenzione dell'Aja del 1981

significa che il problema esiste e persiste e quindi è importante e fondamentale che oggi quest'Assemblea provveda a ratificare una mozione unitaria, sottoscritta da tutti i partiti e senza bandiere politiche.

a volte negli Stati esteri non viene preso in considerazione in quanto è un delitto che prevede una pena edittale fino ad un massimo di quattro anni e quando vengono concesse le attenuanti generiche per tale reato non è possibile procedere ad intercettazioni e svolgere indagini di particolare rilievo. L'impegno da parte del Governo

è che venga costituito un fondo per il gratuito patrocinio in favore delle famiglie. Molto spesso i minori vengono portati all'estero, sottratti all'uno o all'altro genitore, perché inizia una separazione consensuale o giudiziale e, nel corso della separazione, il genitore che pensa di essere affidatario del bambino scappa con lui.

di conseguenza, non agevolano in alcun modo il rientro del minore. Perché abbiamo voluto discutere queste mozioni oggi e nella scorsa seduta? Vorrei raccontarvi una delle tante storie che ci hanno indotto a farlo: mi riferisco alla storia di Rebecca e di suo padre. Rebecca ha dodici anni e da quando ne aveva otto suo padre non sa nulla di lei. Quattro anni fa la madre è riuscita a portarla via dalla comunità protetta in cui si trovava e a riportarla illegalmente in Bielorussia, dove la bambina è letteralmente sparita. A nulla sono valsi i provvedimenti giudiziari della giustizia italiana, compresi quelli che hanno condannato penalmente la madre. A nulla sono valsi i processi, gli appelli, le cause, i viaggi, le richieste e le suppliche del padre. un padre che, tranne un fuggevole contatto su un *social*, subito chiuso, non sa cosa sia accaduto a sua figlia e non riesce più nemmeno a ottenere il visto per entrare in Bielorussia, dove la madre l'ha portata e la nasconde.

Ecco perché questo ordine del giorno unitario, che diversamente dai costumi di questo Parlamento, è molto concreto nei suoi impegni e, in particolare, in quelli che rivolge al Governo, ha finalmente lo scopo di dare un percorso, una sicurezza e una protezione a quei genitori ai quali forse toglie definitivamente l'isolamento. I colleghi poco fa hanno già parlato dei punti che sono stati evidenziati nell'ordine del giorno. Vorrei ricordarne in particolare uno: la richiesta che il tema dei bambini contesi o sottratti accompagni l'agenda del Governo ogni qual volta questo si reca all'estero; ogni qualvolta un nostro rappresentante debba, per ragioni collegate al suo mandato istituzionale, avere contatti con quel Paese. È anche attraverso la forza del nostro Paese che quei bambini italiani potranno tornare a casa. Dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico.

Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la legge di stabilità 2016 al comma 74 dell'articolo 1 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali del 50 per le ristrutturazioni edilizie e acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ e la detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, il cosiddetto ecobonus. Tale provvedimento è il frutto di una norma nata nel 2006 e prorogata annualmente dal Parlamento che, a seconda delle necessità contingenti, l'ha modificata fino ad arrivare alla formulazione attuale che ne ha esteso i settori di applicabilità e i contributi erogati. È chiaro ed evidente che ciò non ha permesso ai cittadini di pianificare queste spese così ingenti nel *budget* familiare, obbligandoli a rincorrere di volta in volta le detrazioni del momento. Oggi siamo punto e a capo: a fine anno i benefici per taluni settori si azzereranno e per altri rimarranno in essere in forma estremamente ridotta. Serve stabilizzare gli interventi di Stato, affinché le imprese e le famiglie possano avere un orizzonte temporale di più ampio respiro, così da programmare le spese. Ciò rappresenterebbe una certezza anche per l'economia, che non progredirebbe più a singhiozzo, ma seguendo un percorso di crescita lineare. In tale contesto, vorrei ricordare a tutti gli astanti che un provvedimento di totale rottura e di contrasto alla crisi è stato il piano casa del Governo Berlusconi, dapprima criticato e riprovato dalla sinistra, ma poi adottato e prorogato fino al 2015 dalla totalità delle Regioni, anche quelle di sinistra, in virtù dei suoi effetti benefici, che ha permesso di spianare la strada all'ecobonus. i dati dimostrano come la totalità dei comparti coinvolti ne abbia beneficiato, riuscendo a rispondere efficacemente agli effetti della crisi.

per il recupero edilizio e dell'ecobonus 65 per cento per la riqualificazione energetica, dal 2008 al 2015: - gli incentivi hanno riguardato oltre 12,5 milioni di interventi, e attivato investimenti per 207 miliardi di euro, di cui 178 miliardi di euro hanno riguardato il recupero edilizio e 30 miliardi di euro la riqualificazione energetica. Il valore più elevato nell'intero periodo di applicazione degli incentivi è stato registrato nel 2014, con investimenti nell'edilizia pari a 28,5 miliardi di euro e 1,9 miliardi di euro nei mobili. Per quanto riguarda il settore dei grandi elettrodomestici, la spinta positiva degli incentivi introdotti dall'ecobonus ha permesso, nel 2014, una crescita del settore pari al 3,7 per cento e dell'8,3 Sono questi i dati che scaturiscono da provvedimenti davvero efficaci e non da un misero zero virgola qualcosa. Si tratta di provvedimenti convenienti per l'intero sistema, che smuovono investimenti, creano occupazione, contrastano l'evasione e creano introiti per lo Stato. Introiti, che, come al solito, il Governo Renzi - quello che secondo la propaganda abbassa le tasse ha incrementato nel 2015, non solo grazie all'ampliamento del raggio di applicazione, ma soprattutto a causa dell'aumento dal 4 all'8 per cento della ritenuta d'acconto, fortunatamente senza intaccare il numero degli interventi degli italiani. Ebbene, le misure temporanee non bastano più: è necessaria una politica lungimirante, un programma di incentivi strutturati che permetta agli italiani e alle imprese una pianificazione efficace degli interventi finalizzati a garantire un maggiore sostegno alla crescita della nostra economia, ma soprattutto al miglioramento dell'efficientamento energetico e della tutela del nostro clima, riservando una particolare attenzione alla strategia di ricerca e innovazione nel settore dell'energia, in cui si stima un volume d'affari medio annuo di circa 5,2 miliardi di euro. A tale scopo, naturalmente, non si può prescindere dalle conclusioni della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici in cui sia l'Unione europea che l'Italia si sono poste degli impegni importanti per il 2030, prevedendo il taglio di almeno il 40 per cento delle emissioni rispetto al 1990 e l'incremento dei 27 per cento dell'efficienza energetica. Certamente l'Italia ha fatto molto e non è lontana dagli obiettivi prefissati. Tuttavia questo non basta: è necessario continuare su questa strada, prestando attenzione anche a quanto evidenziato dalla Commissione europea, che delinea un quadro a tinte fosche per il nostro Paese, in cui di produzione nazionale registra valori più bassi rispetto alla media europea; il *mix* energetico differisce da quello dell'Unione europea a 28 Paesi, con una più ampia percentuale di gas e l'assenza del nucleare; la dipendenza da combustibili solidi è superiore rispetto all'Unione europea a 28 Paesi; i prezzi dell'energia elettrica al dettaglio per l'utenza domestica sono in generale sopra la media

del 75 per cento del patrimonio immobiliare è caratterizzato da bassa o bassissima efficienza energetica. Quelli appena esposti sono dati preoccupanti, che descrivono un Paese incapace di competere alla pari con i suoi vicini e tanto meno con le economie più avanzate. È arrivato il momento di colmare questo *gap* e soprattutto di non farsi dare i compiti a casa dall'Europa. È ora che il Governo si impegni ad utilizzare efficacemente sia le risorse economiche che gli strumenti a propria disposizione per creare un Paese più competitivo. Ciò nonostante sono consapevole che l'efficienza e l'efficacia non siano proprio nel DNA di questo Esecutivo, come dimostrano le tre tornate elettorali che quest'anno impegneranno gli elettori italiani. In merito al cosiddetto *referendum* sulle trivelle, permettetemi di manifestare la mia incredulità dinanzi ad una battaglia prevalentemente ideologica intavolata da alcune fazioni politiche che, da una parte, si dichiarano contro la produzione di energia derivante da combustibili fossili, ma poi cercano di bloccare sette miliardi di investimenti, per non considerare le ricadute su occupazione e indotto, indirizzati proprio alla produzione di gas che garantirebbe quella differenziazione delle fonti energetiche per cui il nostro Paese si è impegnato proprio a Parigi. Per tali motivazioni, con la mozione a mia prima firma, impegniamo il Governo a valutare, sin dal Documento di economia e finanza, di rendere permanente la detrazione fiscale al 65 per cento delle spese sostenute per la per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quale forma di incentivazione per la realizzazione di interventi pluriennali; ad effettuare una ricognizione di tutte le forme di sostegno (detrazioni fiscali, certificati bianchi, contributi in conto capitale, contributi della programmazione europea e altri profili di incentivo), al fine di gestire eventuali sovrapposizioni delle tipologie di intervento. Ho quasi terminato, signora 4) ad individuare tipologie di intervento *standard* per il contenimento delle emissioni e il risparmio energetico, stabilendo premialità basate sul rapporto tra costi e benefici, con particolare attenzione ai lavori che colleghino l'installazione di dispositivi elettronici di controllo dei consumi a semplificare la disciplina di regolazione delle attività delle *energy service company*; a trasmettere una relazione annuale alle Commissioni competenti delle Camere. con la speranza che, almeno per una volta, questo Esecutivo vorrà distaccarsi dalle solite contrapposizioni maggioranza-opposizione e non agisca solo per il proprio tornaconto, e voglia accogliere le nostre proposte

Signora Presidente, colleghi, oggi devo parlare, ma avrei voluto rimanere in silenzio. Oggi finalmente si discute di una misura strutturale, che consentirà di mettere i cittadini in condizione di migliorare la loro bolletta energetica. Ricordiamo che, fatto 100 il fabbisogno complessivo di energia in Italia, il 40 per cento viene impiegato proprio dagli edifici, che mediamente ne sprecano ben il 60

mentre qui stiamo parlando di una misura che ci consentirebbe di ridurre del 15-20 per cento la nostra dipendenza dalle importazioni di energia dall'estero. Se qualcuno ha dei dubbi sulle misure e sull'efficienza, ricordo che i consumi di gas si sono ridotti del 22,4 per cento rispetto al 2005, e quelli di petrolio addirittura del 38 quindi, l'efficienza è il nostro vero giacimento petrolifero. Altro che trivelle a mare! Finalmente discutiamo di una misura strutturale sulla salute. Ricordiamo tutti l'emergenza *smog* di qualche mese fa; ricordiamo che la causa principale di inquinamento, di *smog*, per il quale paghiamo un tributo di 80.000 morti all'anno, è proprio la climatizzazione degli edifici; edifici; al secondo posto l'incidenza delle industrie e al terzo quella del traffico. Però, chissà perché, quando si è in emergenza *smog* si pensa sempre a ridurre o a bloccare il traffico. Finalmente questa è una misura che non è l'ennesimo favore alle *lobby* dominanti, a poche, grandi, grandissime imprese. Viceversa, è una misura che può valorizzare due intere filiere e centinaia di migliaia di posti di lavoro: la filiera dell'efficienza e, naturalmente, la filiera di produzione da fonti rinnovabili, che attualmente sono agonizzanti. Quindi, parliamo finalmente di nuovi posti di lavoro; parliamone perché abbiamo anche in questo caso i numeri precisi. Lo studio del CRESME nel 2014 ha confermato che sono stati creati, grazie ad un ecobonus - nonostante sia a singhiozzo 283.000 posti di lavoro diretti e 424.000 con l'indotto. Ricordiamo ancora una volta il dato previsionale fornito dall'accordo tra Confindustria e i sindacati, che parla addirittura di oltre 1,5 milioni di posti di lavoro. Quindi, finalmente parliamo di una misura di politica industriale di medio periodo; una politica industriale - questa sconosciuta

dall'industriale all'edilizia civile, a quella pubblica; riconversione energetica con il passaggio dalle fonti fossili alle rinnovabili; riconversione ambientale, con una gestione più efficiente del patrimonio agroforestale; riconversione del petrolchimico, con passaggio graduale ad una chimica verde vera, pulita e realmente sostenibile; riconversione dei siti inquinati tramite le bonifiche e riconversione del concetto stesso di rifiuto, della tipologia di rifiuti che devono diventare materie prime secondarie: tutte misure che, sommate tra di loro, creerebbero sicuramente ben più di un milione di posti di lavoro. invece siamo a ricordare, come abbiamo fatto il mese scorso, che quest'anno la fiera del Solarexpo non si terrà, dopo diciassette anni, e questo dà la misura di quanto queste filiere siano agonizzanti. Siamo a ricordare che oggi, con una mano promettiamo (con questa mozione), mentre da diverso tempo togliamo con l'altra mano. Abbiamo tolto parecchio a queste filiere con la riforma sugli oneri in bolletta; riforma che ha ribaltato il concetto della progressività e che ha, quindi, scoraggiato tutti gli interventi di efficientamento energetico e di autoconsumo presenti e futuri. A che *pro*? Qualcuno va negli *States* a farsi bello, a far vedere un bellissimo esempio di centrale a fonti rinnovabili quando qui da noi andiamo nella direzione opposta: opposta: facciamo questa riforma degli oneri; facciamo la riforma dei certificati bianchi, che non sosterrà più gli interventi di efficientamento energetico di piccola entità, rivolti soprattutto all'edilizia; facciamo un nuovo conto termico che non risolve i problemi di quello vecchio e continua a lasciare inutilizzate le risorse stanziate. torniamo invece a vedere cosa comporterebbe la stabilizzazione, dal momento che noi abbiamo 18 milioni di abitazioni in Italia che necessitano di un intervento di manutenzione e che si trovano, fortunatamente dal punto di vista lavorativo, da Nord a Sud. permetterebbe, quindi, a 14 milioni di famiglie che vivono nei condomini, di dimezzare la propria bolletta energetica, di ridurla sensibilmente.

esame è una misura che mette d'accordo tutto il parlamento, dal momento che le mozioni presentate arrivano un po' da tutto l'arco parlamentare. La mia è stata la prima presentata in materia ed non solo dai miei colleghi ma, un po' a macchia di leopardo, anche da molti altri rappresentanti dell'arco parlamentare. anche dalla dichiarazione del partito di maggioranza, viene descritta esplicitamente come una misura *win-win*, quindi non occorre essere grandi esperti di inglese per capire che è una mozione che non comporterà perdite Cos'altro possiamo aggiungere? È da approvare al più presto ed è necessario vigilare affinché il Governo la concretizzi immediatamente, inserendola nel primo atto legislativo utile. L'Italia non può permettersi di aspettare ancora: forniamola finalmente di una misura di politica industriale di medio periodo alla quale le nostre aziende sapranno immediatamente rispondere, dal momento che, se interpellate, tutte rispondono che la prima misura di cui hanno bisogno è la stabilità per poter tornare a programmare gli investimenti. Quindi le aziende potranno tornare a programmare gli investimenti, le famiglie e le imprese potranno tornare a programmare le loro operazioni di efficientamento. Ricordiamo che anche una nota società di studi ha dichiarato che sono misure che si ripagano molto velocemente, addirittura ha calcolato in sette anni, quindi sono misure che si ripagherebbero e poi darebbero un risparmio molto molto sostanzioso (in questo caso la Nomisma lo calcola in 15 miliardi all'anno solo per i due milioni di edifici più vecchi). noi abbiamo aspettato due anni per arrivare a questa mozione e ci auguriamo che, dal momento che in una notte è stato approvato l'emendamento *pro* Total (un emendamento che favoriva una sola singola azienda), azienda), questa misura, nel caso sia inserita come emendamento nel primo provvedimento legislativo utile, sia approvata in maniera ugualmente celere, anche perché questa volta non si favorirebbe un'unica grande impresa ma milioni di normali cittadini e imprese. Non aggiungiamo altro e procediamo il più speditamente possibile. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo di scienze umane «Vito Fornari» di Molfetta, in provincia di Bari. Benvenute e benvenuti al Senato.

voglio svolgere anch'io qualche considerazione senza altre divagazioni su tutto lo scibile che riguarda l'energia nel nostro Paese ma provando a stare

per cento dell'investimento effettuato, rappresentano un significativo volano per la crescita del prodotto interno lordo, per il sostegno di importanti settori produttivi, a partire da quello edilizio, e per il raggiungimento di più elevati livelli di risparmio energetico nel Paese; cioè l'ecobonus. I più recenti dati di analisi sull'efficacia dell'ecobonus, elaborati dal CRESME in collaborazione con la Camera dei deputati e pubblicati lo scorso evidenziano l'impatto positivo nel corso degli anni di tale agevolazione sulla crescita economica grazie alla sua notevole efficacia occupazionale, proprio nel momento di più forte crisi del settore edilizio. Gli incentivi dell'ecobonus, sommati agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, hanno generato nel solo anno 2014 investimenti per un ammontare complessivo di 28,5 miliardi di euro,

alla riqualificazione energetica. I lavori incentivati nel periodo gennaio-agosto 2015 sono stati pari a 15,9 miliardi di euro, che, seppure in leggera flessione rispetto al 2014, rappresentano comunque un dato di notevole importanza. Ma già i primi dati dell'inizio del 2016 sono molto più confortanti e positivi rispetto al 2015. I benefici generati dall'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici e degli incentivi per la ristrutturazione edilizia ovviamente si riflettono positivamente anche sull'occupazione. secondo le stime del CRESME, gli investimenti attivati da tali agevolazioni sono valsi, nel periodo 2011-2015, un assorbimento di 1.163.255 occupati diretti, corrispondenti a una media annua nel periodo di quasi 233.000 occupati; nel solo 2014, 283.200 posti di lavoro diretti nel settore dell'edilizia e 424.800 occupati totali, compreso l'indotto; mentre nel 2015, gli occupati diretti rilevati sono stati 234.000.

1.128.000 occupati totali. gli investimenti che si sarebbero persi, senza sgravi irpef, sarebbero stati pari a 15,9 miliardi di euro su un totale di 28,4 miliardi, mentre la perdita in termini di occupazione sarebbe ammontata a 158.591 posti di lavoro; se si prende a riferimento un periodo più ampio che va dal 2011 al 2014, la mancata attuazione delle agevolazioni avrebbe comportato la perdita di 47,1 miliardi di investimenti e gli effetti sull'occupazione diretta avrebbero comportato una riduzione di 468.769 posti di lavoro;

2014. Vorrei concentrare l'attenzione di quest'Aula anche sui benefici in termini ambientali dovuti alla presenza dell'ecobonus. Il rapporto annuale 2015 sull'efficienza energetica, curato dell'ENEA sulla base dei dati disponibili al 30 aprile 2015, ha evidenziato gli effetti positivi dell'ecobonus in termini di risparmio energetico e di impatto positivo sull'ambiente. Nel periodo che va dal 2007 al 2013, l'ENEA ha calcolato un risparmio di energia primaria pari a 0,913 megatep, equivalenti ad oltre 9.900 gigawatt orari per anno di energia finale, di cui oltre 1.650 gigawatt orari per anno derivanti da interventi incentivanti nel 2013. Tali dati evidenziano il notevole impatto in termini di risparmio energetico e di minori emissioni inquinanti nell'ambiente, che possono derivare dall'attuazione di interventi, come la schermatura degli edifici, il cambio degli infissi e l'utilizzo di impianti di riscaldamento efficiente e tecnologicamente avanzati. L'efficienza energetica ha quindi assunto negli anni una rilevanza sempre maggiore e costituisce la principale chiave di sviluppo per nuovi modelli operativi in un'economia globalizzata. Perciò, investire sul risparmio energetico negli edifici e su modelli di reti intelligenti è fondamentale per un nuovo sviluppo economico del Paese. Una politica di risparmio energetico sul patrimonio edilizio italiano, attivata su 12 milioni di edifici, è in grado di generare risorse economiche private, mettendo a reddito gli oltre 20 miliardi annui di energia che invece viene sprecata.

Costruire edifici sempre più abitabili, che possano migliorare la qualità della vita dei loro occupanti e integrarsi all'ambiente circostante, alla luce di ottime *performance* ambientali e di una riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, aiutano il *business* della filiera edilizia, anziché affossarlo. Proprio oggi - è importante ricordarlo - si è aperto un importante salone, quello del mobile a Milano, che parla già da tempo questo linguaggio. Ed è per questa ragione che la mozione del Partito Democratico chiede sostanzialmente chiede sostanzialmente di dare stabilità, a decorrere dall'anno 2017 all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici. La stabilizzazione di questa agevolazione rappresenta una scelta di politica industriale che incontrerebbe il favore sia del sistema economico sia dei contribuenti (come abbiamo visto dai dati). un rallentamento e gli ordinativi hanno iniziato a diminuire in modo deciso. È del tutto evidente che la mancanza di certezze sulla defiscalizzazione dei futuri investimenti di efficientamento rappresenta un freno alle decisioni di investimento dei contribuenti. inoltre di inserire l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici all'interno di un complesso quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali, avendo cura di garantire in ogni caso un effettivo vantaggio agli interventi volti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del patrimonio, tenendo fermo a tal fine l'attuale parametro normativo che prevede una differenza di 15 punti tra la predetta agevolazione (il cosiddetto ecobonus) e quella riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione. Chiediamo poi di considerare la possibilità di rimodulare i tempi dell'erogazione dell'incentivo, tempi che potrebbero essere non fissi, ma crescenti con l'ammontare della spesa, al fine di rendere conveniente la detrazione fiscale anche per microinterventi.

la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (come già si è iniziato a fare con legge di stabilità 2016) e di edifici di proprietà di ONLUS, la riqualificazione di edifici interi, il consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree a rischio sismico, nonché il consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali, ivi comprese le strutture alberghiere e ricettive in generale. Infine, chiediamo di estendere l'applicazione dell'agevolazione alla costruzione di nuovi edifici, nel caso siano rigorosamente seguiti i criteri di bioedilizia

in modo che queste agevolazioni possano rappresentare davvero un volano importante di sviluppo, com'è avvenuto negli anni precedenti.

Signora Presidente, siamo arrivati finalmente a discutere di queste mozioni. Era un po' di tempo che ci eravamo impegnati per cercare di capire in che termini una stabilizzazione degli ecobonus potesse mettere questo

della capacità imprenditoriale di un Paese che ha visto scemare nel tempo quella che era una *green economy* che ha funzionato molto bene negli anni passati. Era anche chiaro che, di fronte al al perdurare della crisi economica, gli investimenti in edilizia, in risparmio energetico, in fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca e, più in generale, nella *green economy* possono e devono rappresentare un'importante occasione per ridare slancio all'economia italiana, permettendo di coniugare l'obiettivo di una maggiore competitività e modernizzazione del Paese con la necessità di adottare modelli di sviluppo maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale. Caratterizzante la XVII legislatura è stata anche la conferma in diverse occasioni, non ultimo nell'ambito dell'esame del cosiddetto allegato Kyoto al Documento di economia e finanza del 2015, del percorso verso un'economia a basso contenuto di anidride carbonica, che per l'Italia risulta fondamentale ai fini del raggiungimento degli impegni presi a livello internazionale ed europeo. Ed è proprio a livello europeo che l'adozione del pacchetto clima ed energia ha dato risultati positivi sul versante del rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto; noi siamo tra i Paesi che li hanno raggiunti per primi e le ultime statistiche annuali di Eurostat evidenziano la continuità della tendenza positiva: nel 2013 nell'Unione europea le emissioni di anidride carbonica derivate dalla combustione di combustibile fossile sono diminuite del 2,5 per cento rispetto al 2012 e il nostro Paese ha dato una mano per raggiungere questo risultato. Il Consiglio europeo del 22 e 23 ottobre 2014 ha raggiunto l'accordo quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030. Anche in questo caso già nella passata legislatura ci siamo messi in moto con una serie di provvedimenti che hanno permesso al nostro Paese di essere un po' all'avanguardia, ma poi abbiamo visto scemare il tutto con una serie di provvedimenti che hanno caratterizzato la prima parte della della XVII legislatura, quando alcune azioni di carattere normativo non hanno messo il comparto in condizione di eccellere come succedeva prima. Nel 2014 con il decreto legislativo n. 102 si sancisce il ruolo fondamentale dell'efficienza energetica come strumento strategico nell'attuale scenario europeo per affrontare sfide come come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, il rilancio della crescita economica, la creazione di nuovi posti di lavoro e l'aumento della competitività delle aziende intervenendo in diversi settori ritenuti in grado di cogliere le opportunità offerte dal risparmio energetico, dall'edilizia ai trasporti passando per le produzioni. casca l'asino, perché tutti questi passaggi che si erano potenzialmente previsti e stabilizzati anche solo per poco tempo hanno visto calare di colpo le loro capacità di

sicuramente dovevamo adottare iniziative volte a garantire la definizione di un quadro normativo certo ed esaustivo a tutela degli investimenti nel settore delle rinnovabili, sia per ridurre le dipendenze dalle importazioni di energia sia per tutelare le legittime aspettative delle non è stato proprio fatto, signora Presidente, anche tenendo conto degli effetti positivi sull'economia e sull'occupazione, dato che nel solo comparto delle energie rinnovabili le imprese dell'Unione europea sviluppano un fatturato di 129 miliardi di euro e danno lavoro a più di un milione di addetti. Per raggiungere questi obiettivi è stato necessario effettuare operazioni dirette alle piccole e medie imprese, al rilancio del settore degli investimenti e dell'edilizia, al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e dei processi produttivi, allo snellimento e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione degli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili. Erano obiettivi strategici sicuramente da prendere in considerazione; assumono oggi come non mai importanza per il rilancio degli investimenti in innovazione tecnologica e la riduzione dei consumi energetici e l'incremento dell'efficienza ma sembrano a questo punto discretamente in dubbio.

con effetti positivi sul bilancio del Paese, in quanto non solo rappresenta un importante sostegno al rilancio dei consumi, ma contribuisce anche all'emersione del sommerso in settori ritenuti strategici per la ripresa economica, come quello edile; il nostro Paese vanta inoltre una il nostro Paese vanta inoltre una fiorente industria in diversi settori strettamente correlati all'efficienza energetica. Negli ultimi anni si è assistito ad una consistente crescita dei sistemi di accumulo di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla fonte solare, i quali hanno dato vita ad un mercato nel quale l'Italia è all'avanguardia con numerose aziende *leader* a livello Partendo da tutte queste considerazioni, il comparto abitativo ha un ruolo di fondamentale importanza nelle nelle politiche per l'efficienza energetica sicuramente strategico, visto che agli immobili è ascrivibile circa il 36 per cento del consumo complessivo di energia; pertanto, si vincola il Governo a rendere permanenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio, questa norma che riguarda la questione incentivi. Noi abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi di far sì che quest'Aula potesse votare una mozione che mettesse in condizioni un comparto di riprendersi e di stabilizzarsi e di far sì che gli investimenti siano certi

calo drastico dei dipendenti e, quindi, dell'occupazione. Solamente nell'eolico si calcolano circa 4.000 soggetti che hanno perso il posto di lavoro. chiediamo a voce alta e cerchiamo di spronare il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere finanziario, volta alla stabilizzazione normativa delle attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; e, nel contempo, a reperire le opportune risorse finanziarie da indirizzare a sostegno di misure per la riduzione del numero di rate annuali relative al recupero delle spese sostenute dai contribuenti

ad incentivare, nell'ambito delle politiche finalizzate alla maggiore crescita delle fonti energetiche rinnovabili, la realizzazione di sistemi di accumulo a batterie installati all'interno di edifici in abbinamento

di fare retromarcia e anche un *mea culpa*, mettendo in condizione anche chi mi sta ascoltando dai banchi del Governo di ragionare con serenità per quanto riguarda un argomento, quello delle energie, che mai come in questo periodo è assolutamente di primaria

Signora Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, se avessimo l'abitudine di dedicarci un po' di più e un po' meglio alla misurazione della qualità della produzione legislativa, probabilmente otterremmo un miglioramento sostanziale della qualità stessa delle nostre leggi, nella consapevolezza che fare delle buone leggi rappresenta di per se stesso un prerequisito per il funzionamento di uno Stato democratico e rappresenta anche un buon metodo per recuperare il rapporto fra la piazza e il palazzo, dopo che un grave cortocircuito lo ha irrimediabilmente mortificato. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e che a supporto di una completa e precisa illustrazione delle varie mozioni sull'argomento di nostro interesse hanno portato dati puntuali, che confermano come e quanto

di una politica di sviluppo del comparto edilizio e, al tempo stesso, di un'attività per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera abbia presentato un esito assolutamente positivo, con benefici dal punto di vista economico. È infatti accertato che il saldo economico tra i benefici erogati e gli introiti fiscali (IRPEF, IVA ed IRES) è stato significativamente positivo. Ma non sono stati importanti

alla riduzione della emissione di CO2 in atmosfera con evidenti riflessi positivi sulla salute della popolazione. effettuati in questi anni sono stati misurati in 207 miliardi circa, 178 per il recupero edilizio e 30 per la riqualificazione energetica. Complessivamente, si parla di oltre 12,5 milioni di euro di interventi che hanno prodotto beneficio per l'occupazione. Gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica hanno determinato due milioni di occupati nel periodo 2008-2015 questa considerazione appare tanto più rilevante quanto più si consideri il periodo particolarmente delicato per gli aspetti della crisi, che si è giovato certamente di una spinta energica sul versante dell'occupazione. Questi dati sono detti in modo chiaro ed incontrovertibile nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione ambiente qui in Senato (ma anche alla Camera). La documentazione prodotta - mi riferisco a quella del CRESME, della Confartigianato e della Confindustria Confindustria - e gli elaborati degli Uffici studi sia della Camera che del Senato hanno confermato che il periodo preso in esame, calcolando i minori introiti legati agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e, dall'altro, considerando la quota di gettito per lo Stato derivante dai consumi e dagli investimenti investimenti determinati dai redditi aggiuntivi ai nuovi occupati, ha determinato un saldo positivo per lo Stato di circa 10,5 miliardi di euro, che potrebbero salire a poco più di 15 miliardi di euro ricomprendendo gli effetti indotti a beneficio delle famiglie e delle imprese. LETTIERI). Credo che questi dati siano incoraggianti e debbano spingere il Governo a fare ciò che si chiede con la mozione che Conservatori e riformisti pongono

Sostanzialmente, riteniamo necessario superare la fase della contingenza, che porta prevalentemente a prorogare

Un altro aspetto per il quale vogliamo impegnare il Governo e che riteniamo sia in perfetta sinergia con le misure fiscali e il recupero del 65 per cento delle spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico degli edifici edifici riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per i contratti di servizio energia destinati all'uso domestico. su tali contratti permane l'incertezza che si è venuta a creare tra gli operatori in tema di aliquota IVA da applicare. Alcuni soggetti pubblici

favorendo un'interpretazione univoca della norma. Peraltro, voglio ricordare che anche alla Camera dei deputati il problema che ho testé esposto è stato illustrato, fino a diventare un punto cogente di richiesta entrato in un ordine del giorno, essendosi previsto nell'ambito del decreto legislativo di attuazione della direttiva

e comunque uniforme. Appare pertanto logico che, ove sia applicata l'aliquota agevolata del 10 per cento per le pubbliche amministrazioni, tale misura

Queste sono le richieste che avanziamo al Governo. In considerazione della ragionevolezza che esse contengono in termini di compatibilità con il il bilancio dello Stato, ma anche nella consapevolezza dei dati che ho illustrato (sulla cui attendibilità richiamo il Governo a fare le valutazioni in ordine ai documenti depositati in modo ufficiale presso le competenti Commissioni), credo che vi siano tutte le motivazioni perché il Governo possa esprimere il proprio benevolo parere mostrando un'adeguata attenzione a sostegno dell'economia, ma anche della coesione sociale e del miglioramento dei livelli di tutela della salute nel nostro Paese.

le misure di agevolazione per la riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia degli edifici, a distanza di anni dalla loro entrata in vigore, non sembrano rappresentare un costo per le finanze pubbliche. Anzi, i calcoli effettuati dal CRESME evidenziano come l'applicazione degli ecobonus e delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie abbiano generato, nell'intero periodo di riferimento, che va dal 1998 ad oggi,

Con il comma 87 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), si sono estese le detrazioni per l'ecobonus del 65 per cento anche agli «Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati», riconoscendo l'importanza strategica e l'alta valenza sociale degli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia effettuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica. la formulazione utilizzata dal legislatore per indicare i soggetti che intervengono su detto patrimonio non indica (come invece è riportato ai successivi commi 89 e 90 in materia fiscale) anche gli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi per le case popolari, ma istituiti nella forma di società e rispondenti ai requisiti della legislazione della Comunità europea in materia di *in house providing* e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. La suddetta formulazione, per così dire monca, non può e non deve penalizzare soggetti che gestiscono e intervengono sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica per il mero fatto di essere istituiti in forma di società. Per quanto concerne il conto termico, il sistema già prevede premialità per interventi globali sull'edificio e in caso di *deep innovation*, ma sarebbe opportuno prevedere ulteriori premialità in caso di interventi su edifici storici o in caso di applicazione di protocolli energetico-ambientali, che non considerino solo la riduzione dei consumi energetici, ma anche, in senso più ampio, l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e il risparmio di altre risorse, quali, ad esempio, l'acqua o il terreno (ad esempio sistemi LEED, sistemi GBC o similari). La normativa vigente prevede infine la possibilità di detrarre gli interessi per i mutui contratti per costruire o ristrutturare la prima casa solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia rivolti a trasformare gli edifici, escludendo gli interventi di restauro e risanamento conservativo, riservati, ad esempio, agli immobili vincolati, che che pure sono quelli più costosi e più delicati. Sulla base di tutto questo, con la mozione si chiede un impegno da parte del Governo per: dare stabilità, a decorrere dall'anno 2016, all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici; ricomprendere, fra gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, che possono usufruire dell'agevolazione fiscale del 65 per cento per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, anche gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società

chiesti in questa mozione sono vasti. Ne ho approfittato per inserire tutta una serie di richieste che provengono anche dal territorio e che, se assecondate, darebbero ulteriore impulso agli interventi di riqualificazione energetica e, soprattutto, migliorerebbero la qualità energetica dei nostri edifici. Fra questi, chiederei al Governo di prestare un'attenzione particolare per ricomprendere tra gli istituti autonomi per le case popolari anche quelli costituiti in forma di società perché si tratta di un caso unico e assolutamente minimale all'interno del panorama

all'emersione del sommerso - e credo ci portino ad avere un'attenzione particolare. Mi auguro pertanto che il Governo possa cogliere queste sensibilità che ho illustrato nella mia mozione.

gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto hanno già opportunamente sottolineato l'importanza degli ecobonus edilizi nel quadro della politica energetica, ambientale ed economica dei Governi succeduti dal 2007 ad oggi. La discussione parlamentare di oggi, ancorché tardiva, è un'importante opportunità per ragionare sui diversi punti da segnalare al Governo, anche in vista delle legge di stabilità e di bilancio per il 2017. Entrando più nello specifico, vorrei qui sottolineare alcuni punti della mozione n. 456, a firma di molti senatori del Partito Democratico, alcuni dei quali, peraltro, si rinvengono anche nelle altre mozioni sullo stesso tema, auspicando approvazioni trasversali e il più possibile condivise. Il primo punto è la richiesta di stabilizzare l'ecobonus, o almeno di provvedere a una sua proroga pluriennale, in modo da farlo entrare più stabilmente nel sistema fiscale nazionale. È vero che uno stanziamento annuale ha il tendenziale vantaggio di spingere gli utenti ad accelerare i tempi dei lavori. Tuttavia, gli interventi complessi sui grandi edifici - ossia proprio quelli di maggiore efficacia in termini di risparmio energetico - spesso non riescono a esaurirsi nel corso di un anno e, quindi, sfuggono alla possibilità di accedere con modalità semplice all'incentivo. In secondo luogo, andrebbero rivisti i tempi di erogazione dell'incentivo, che potrebbero non essere fissi ‑ ora sono di dieci anni ma crescenti con l'ammontare della spesa, al fine di rendere più conveniente la detrazione fiscale anche per i micro-interventi. Un terzo punto importante riguarda l'estensione dell'ecobonus, con meccanismi fiscali da definire, anche a soggetti diversi dalle famiglie e dagli edifici di edilizia residenziale pubblica. Infatti, l'efficienza energetica è oggi particolarmente deficitaria anche per altri edifici, come - ad esempio - per quelli di proprietà di enti *no profit*. Anche se interventi di questo tipo non potrebbero utilizzare in modo diretto la leva fiscale, il loro costo nel medio periodo sarebbe nullo, come sottolineato da molti interventi. L'ecobonus potrebbe, inoltre, essere esteso anche alla costruzione di edifici nuovi, quando siano rigorosamente seguiti criteri di bioedilizia o di di energia zero o quasi zero, specialmente se essi vengono costruiti in sostituzione della cubatura di edifici esistenti a scarsa efficienza energetica. Infine, è fondamentale organizzare studi indipendenti più sistematici sull'efficacia di questa misura fiscale, che ne mettano bene in evidenza i vantaggi, oltre gli eventuali svantaggi, adottando diversi punti di vista. Auspico, dunque, che in un prossimo provvedimento legislativo l'ecobonus venga meglio articolato e segmentato, sfruttando così in misura maggiore le spinte economiche e ambientali che possono derivare da tale misura. È impressione condivisa che l'ecobonus sia stato uno degli interventi fiscali più importanti e vincenti dell'ultimo decennio di Governo. Tra le altre cose, esso ha dato ossigeno a molte imprese, in un momento di profonda crisi del comparto edilizio; ha migliorato la qualità della vita e diminuito i costi energetici per molte famiglie; ha permesso enormi risparmi di combustibili fossili: tutti vantaggi conseguiti a costo praticamente nullo. Vale quindi la pena di cesellare meglio questa misura, migliorandola, estendendola e stabilizzandola.

non solo perché sono un convito sostenitore della stabilizzazione dell'ecobonus, ma soprattutto per rimarcare gli effetti che tale iniziativa ha avuto sul sistema italiano di economia reale. Indubbiamente, gli aspetti positivi non sono riassumibili solamente in termini di risparmio energetico, rispetto per l'ambiente e la salute, ma anche per l'effetto indiretto che ha generato sull'economia e l'occupazione, in una fase di congiuntura finanziaria così difficile come quella degli ultimi anni, con un intervento anticiclico di vero stimolo alla economia reale. L'ecobonus ha rappresentato e rappresenta un segnale positivo e - direi molto più concretamente - un sospiro di sollievo per le imprese come per i professionisti: esso rappresenta senza dubbio una misura efficace, che permette di perseguire la strada della riqualificazione energetica, nell'ottica dell'efficienza e del risparmio, stimolando, al contempo, investimenti e crescita. In un momento come quello attuale, dove gli investimenti dei privati nel campo dell'edilizia e dell'impiantistica sono fermi per mancanza di di domanda, gli incentivi statali rischiano di diventare l'unico motore in grado di far veramente ripartire in pieno la nostra economia. È quindi comprensibile che, da più parti, ci sia un appello affinché il Governo mantenga attivo negli anni l'ecobonus per gli interventi volti al conseguimento del risparmio energetico. Basti pensare che la componente della domanda legata alle ristrutturazioni e all'efficienza energetica ha fatto da cuscinetto al pesante ridimensionamento del settore immobiliare dopo la crisi finanziaria del

del patrimonio esistente. Ancora, per completezza, giova ricordare che, dal 2008 al 2015, le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti

periodo 2008-2015, ha riguardato oltre due milioni di occupati, con una media di 111.000 occupati diretti all'anno. Ho premesso tutto questo per ricordare a quest'Assemblea che i provvedimenti giusti, ovvero quelli volti ad accrescere uno sviluppo dell'economia reale, vanno non solo sostenuti, ma anche e soprattutto Penso - e i numeri lo dimostrano - che lo strumento dell'ecobonus non solo porta con sé gli aspetti positivi nella economia interna, ma rappresenta anche un lungimirante adeguamento per quanto riguarda i dettami europei. Proprio in questi giorni si sta aprendo un dibattito sugli sviluppi della strategia quadro per l'Unione dell'energia, la quale mira a integrare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento nelle politiche energetiche dell'Unione stessa, attraverso una serie di interventi volti a eliminare la dispersione energetica degli edifici, a massimizzare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, nonché ad integrare tali sistemi nel sistema dell'energia elettrica e a sostenere l'efficienza energetica nell'industria. Mi chiedo, quindi, quale migliore occasione per promuovere e integrare le politiche europee sull'energia con provvedimenti di stimolo nazionali come questi? La stessa strategia identifica e suggerisce una serie di azioni volte a facilitare la ristrutturazione degli edifici. Ad esempio, si invitano gli Stati membri a rivedere la normativa al fine di trovare un modo di ripartire tra proprietari e inquilini i benefici economici derivanti dall'efficienza energetica. Infatti, nel caso di immobile affittato, è limitato o nullo l'interesse dell'inquilino a investire in una migliore efficienza di un bene non di sua proprietà e altrettanto limitato l'interesse del proprietario a investire in quanto non ne

L'Italia - e lo possiamo dire con una punta di orgoglio - è già sulla buona strada. Le agevolazioni fiscali contenute nei provvedimenti sull'ecobonus vanno proprio in questa direzione. Investire in efficienza energetica vuol dire investire nel futuro, un futuro con aspetti e potenzialità diversi dai decenni scorsi. Il mondo inevitabilmente evolve a ritmi tanto veloci quanto esigenti. Adeguarsi a *standard* europei vuol dire non solamente allinearsi a una strategia, ma anche e soprattutto generare una omogeneità sociale e ambientale comune a tutti i cittadini europei. Concludendo, l'attenzione per l'ambiente, in tutte le sue forme, si esprime come un'attenzione all'edilizia di qualità, che non consumi nuovo territorio ma punti su innovazione, sicurezza e bellezza. Estendere, confermare e rimodulare l'ecobonus non solo significa ridurre i consumi energetici e l'inquinamento, ma rappresenta anche un vantaggio sia per le famiglie che per le casse dello Stato.

e si chiama "zerowatt", ovvero il kilowatt che abbiamo risparmiato. Ci sono costi indiretti, di cui si parla ancora troppo poco e che hanno a che fare con la salute umana, con i cambiamenti climatici, con i costi per le migrazioni ambientali - non solo quelle causate da fame e guerre - che si stanno imponendo proprio per il prelievo delle fonti fossili da quei Paesi. Stiamo oggi analizzando come una felice intuizione che il legislatore italiano ha avuto molti anni fa, ovvero quella di favorire fiscalmente le ristrutturazioni edilizie, abbia trovato la sua strada maestra a partire dal 2006, con una rilevante crescita anche della percentuale di recupero fiscale apportata, qualora si tratti di ristrutturazione con finalità di riduzione dei costi energetici. Da allora si è vista crescere, anno dopo anno, la platea dei soggetti ai quali poter offrire questa opportunità e si è vista implementare la numerosità degli interventi fiscalmente deducibili, ai quali quindi l'ecobonus può essere utilmente applicato. Questo testimonia una cosa indiscutibile, a cui tutti oggi hanno fatto riferimento nell'esplicitare la loro relazione: si tratta di uno strumento valido che procura occupazione; incrementa le imprese attive e la loro qualità tecnologica; rende possibile una riconversione industriale; implementa la stessa ricerca sulle rinnovabili e sulle diverse forme di efficientamento possibili, migliorando quindi la nostra competitività di Paese, riducendo di molto i costi delle famiglie e delle aziende rendendo contestualmente meno grave il *deficit* determinato dalla bilancia dei pagamenti; causa la necessità energetica da fonti fossili del Paese Italia. Se sono veri - e non ne possiamo dubitare - i dati sull'occupazione, va detto che quei 130.000 occupati annuali in più, registrati nel corso di questi anni grazie esclusivamente all'esistenza dell'ecobonus, valgono in termini anche di costo - per mancata Cassa integrazione e mancato valore economico per la disoccupazione - la bellezza di 2,4 miliardi l'anno, che si sommano a tutti i costi - per la verità lo abbiamo già sentito - che sono sulla bilancia dei pagamenti del nostro Paese in positivo, nonostante il valore economico in campo sia gravoso per la deduzione fiscale prevista. inoltre, l'impegno internazionale che ci siamo assunti con la COP 21 di Parigi, che vorremmo diventasse la certificazione della nostra serietà, come Governo italiano e come Parlamento, essendo questo lo strumento principe per raggiungere quell'obiettivo. Sappiamo che si può raggiungere e superare l'80 per cento delle emissioni degli edifici in atmosfera agendo sulle leve del miglioramento tecnologico grazie all'applicazione di coibentanti nei solai e sulle pareti, con la sostituzione di serramenti o degli pareti, con la sostituzione di serramenti o degli elettrodomestici (con il semplice cambio di lampadine o con un banale intervento su caldaie e pompe di calore). Le potenzialità, dunque, sono enormi e probabilmente - come è già accaduto per le rinnovabili - sono ulteriormente suscettibili di positive sorprese future, frutto di ricerche e capacità di innovazione di un mercato sempre più *green* e interessato. L'ambiente ha un costo e si va fuori mercato: tempo fa dicevano gli scettici. Oggi questo non lo esprime quasi più nessuno, anche perché sappiamo che le cause ambientali determinano 84.000 morti in Italia, 400.000 in Europa. E, quindi, il valore assoluto che hanno la sobrietà e la qualità dell'abitare, del muovere e del produrre è diventato la via regina da utilizzare. Stabilizzare, dunque, l'ecobonus fino al 2020 è quanto chiediamo oggi. Bisogna comprendere che l'azione attivata dal 2006 e poi dal 2016 - ricomprendendo anche la sicurezza antisismica - va stabilizzata. Occorre ridurre, laddove è possibile, i dieci anni previsti per l'ammortamento fiscale nella spesa dell'efficientamento; semplificare e ridurre la numerosità delle forme di finanziamento e incentivazione oggi previste sul medesimo intervento, recuperando, laddove è necessario, i fondi su incentivi e sussidi all'uso delle fonti fossili, promuovendo un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che renda i territori più a rischio maggiormente resilienti.

L'intelligenza e la creatività applicata all'efficienza è il nostro nuovo paradigma, come la sfida che dobbiamo cogliere grazie alla volontà univoca del Senato di stabilizzare l'ecobonus.

la legge di stabilità per il 2016 prevede che possano usufruire della detrazione del 65 per cento anche gli istituti autonomi case popolari che, nel 2016, sosterranno spese per interventi sugli immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Alcune mozioni contengono nel dispositivo l'impegno al Governo a fare ciò che è già presente nella legge di stabilità. Inoltre, la legge di stabilità prevede che nei condomini la detrazione degli inquilini incapienti possa essere ceduta alle imprese che realizzano i lavori, in maniera tale che non vada perduta la possibilità di realizzare quella operazione utilizzando l'incentivo. Questa è un'ipotesi - secondo me - poco nota e poco praticata, ma particolarmente interessante, che fa parte della legislazione vigente.

giustamente, sollecitano il Governo a impegnarsi a fare di più introducendo altre forme di agevolazioni per investimenti nelle abitazioni che le rendano ancora più efficienti sotto il profilo energetico

cioè di classe A o B, di nuova costruzione o ristrutturate dalle imprese costruttrici nel corso del 2016. Molte mozioni chiedono di fare qualcosa di simile quando questa previsione è già legislazione vigente.

alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie - spesso si tratta di operazioni che casa per casa, edificio per edificio, vanno assieme nella scelta dei cittadini e negli investimenti delle nostre famiglie - si sta parlando (qui è il vice Ministro dell'economia che parla e non un esperto di ristrutturazioni edilizie e nemmeno di politica energetica, e per fare questo avreste dovuto chiamare un altro vice Ministro, un altro Sottosegretario o un altro Ministro) di detrazioni

dal lontano 1998, quando un relatore alla legge che allora si chiamava finanziaria, allora relativamente giovane e il cui nome non vi rivelo ma che si può trovare, presentò un emendamento per introdurre

di fronte alle argomentazioni sviluppate nelle mozioni che esaltano questa misura, si ingigantisce e raggiunge limiti veramente preoccupanti. Una volta detto questo,

Da allora, e cioè dal 1998 per le ristrutturazioni edilizie, e poi dal 2006 per quanto riguarda l'ecobonus, noi abbiamo avuto interventi di rinnovo sostanzialmente annuale, con modificazioni interne molto significative: il massimo degli investimenti detraibili, il volume della detrazione, il numero degli anni in cui è possibile effettuare la detrazione. Questi sono cambiati, ma non è cambiata la valenza annuale. Perché? È ovvio. Dire che la norma è in vigore con un'agevolazione così intensa solo per un anno spinge in quello stesso anno a concentrare gli investimenti. e che è stato richiamato per ultimo dalla senatrice Puppato. È chiaro che si vuole dare un connotato anticiclico alla misura e, quindi, si capisce la limitazione nel tempo. Dare, però, come limitazione un solo anno, poiché le decisioni più impegnative d'investimento implicano un periodo di tempo e di preparazione e poi di effettuazione più lungo, potrebbe non farle ricadere in positivo sotto l'ombrello della detrazione, a causa di questa limitazione del tempo. Allora, per dirlo chiaramente, io sono venuto qui, questa sera, a nome del Governo per dire quanto segue. Siccome il Governo riconosce fondata questa valutazione, è d'accordo ad accettare l'impegno,

Perché, secondo me, i proponenti potrebbero accettare questa soluzione? Perché decidere oggi, sotto il profilo economico, che un investimento come quello relativo all'ecobonus abbia un orizzonte più che decennale? Dire stabilizzare vuol dire per sempre, ma noi abbiamo degli operatori che hanno bisogno di sapere che nel 2025 ci sarà l'ecobonus? Non escludo che qualche caso ci sia ma, se stiamo parlando degli investitori e delle famiglie, è tendenzialmente vero l'opposto. Se dico oggi che nel 2025 sarà in vigore, temo che quei vantaggi economici, sociali e ambientali, di cui chi ha parlato si occupa occupa e s'intende molto più di me, vengano a non essere conseguiti a causa del rinvio nel tempo dell'investimento. Altra cosa, però, riguarda affrontare il tema della certezza del diritto. Si sa che in un grande condominio, dove si devono mettere assieme tante persone e tante famiglie per fare l'investimento e adire l'agevolazione l'agevolazione - ognuno di noi ha un'esperienza di un'assemblea di condominio, che spesso presenta caratteri di rissosità che la fa somigliare ad assemblee che ci sono più note -

preso atto del risultato positivo conseguito negli anni, dal 1998 ad oggi - sono passati Governi di tutti i colori - attraverso misure di questo tipo, impegna il Governo a stabilizzare l'ecobonus per tre anni.

avanzata da ognuno dei Gruppi con riferimento in particolare alla ristrutturazione degli edifici e così via e anche all'ecobonus, (spesso non del tutto chiaro nel suo rapporto con la misura che si propone), allora è chiaro anche continuare a proporre che le mozioni facciano un gesto politicamente molto impegnativo, che il Governo accetta, e cioè stabilizzare l'ecobonus per tre anni. Non posso, però, fare a meno di dire che non sono in grado di condividere

mozioni, per quanto riguarda il dispositivo chiedo ai proponenti di limitarlo alla seguente frase: «impegna il Governo a dare stabilità, per il triennio 2017-2019, all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici».

piuttosto che sulla politica riguardante lo sviluppo del settore industriale e degli strumenti per il risparmio energetico. Naturalmente sono tutti argomenti di cui non voglio ridurre la portata; al contrario, sto addirittura dicendo che vanno persino un po' al di là delle mie personali personali competenze e, quindi, avrei un'incertezza nel formulare i pareri. Io penso che la cosa che propongo sia talmente semplice, se venisse accettata, ma talmente rilevante sul piano politico che dovrebbe che dovrebbe indurre tutti i proponenti a convergere su di essa. Naturalmente, se non lo faranno, sarò pronto a formulare i mie pareri contrari (molto spesso) o favorevoli sul resto delle mozioni, segmento per segmento, mozione per mozione. che il Senato compia quello che si chiama un atto di indirizzo sul Governo molto significativo, come quello che vi ho proposto. ultima considerazione, non sono invece in grado di accettare, perché il Governo non le condivide, proposte che riguardano una radicale modificazione, in termini di accorciamento, dei tempi di effettivo recupero della detrazione, Proprio i numeri che voi avete citato e il successo straordinario di queste misure dimostrano che il problema non è la durata della detrazione, tanto più in un regime di bassissima inflazione. Quello che conta è essere certi della detrazione e avere il tempo necessario per attivarla attraverso l'investimento, senza l'ossessione della fine dell'anno.

riformulazione: «impegna il Governo a dare stabilità per il triennio 2017-2019 all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici».

Signor Presidente, la valutazione sulla proposta del Governo è stata tempestiva, nel senso di adesione, perché il Senato possa dare un messaggio chiaro e preciso in relazione all'assunzione da parte del Governo di un impegno che riteniamo assolutamente utile per i motivi illustrati nei nostri interventi. Pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Conservatori e Riformisti,

in quella sede sia possibile sollevare anche le altre tematiche, dagli *extra*-*bonus,* agli istituti autonomi per le case popolari, alla semplificazione delle procedure, all'anticipazione delle rate.

Il cosiddetto ecobonus ha un effetto assolutamente positivo dal punto di vista economico, perché ha prodotto moltissimi posti di lavoro e

- questa misura fa davvero bene all'economia, all'ambiente e all'energia. Se avessimo investito tutti i regali fatti alle società petrolifere per incrementare l'ecobonus, credo che oggi avremmo non solo dei grandi miglioramenti ambientali, ma anche posti di lavoro

Le fonti alternative energetiche richiedono infatti ricerca. Per cui, il personale viene impiegato anche in questo. Ci sono questi numerosi aspetti.

il recupero fiscale avviene nell'arco di un periodo lungo (dieci anni). Il mancato beneficio immediato viene compensato da questa durata.

efficientamento degli edifici consente di realizzare molti interventi anche su quelli già esistenti. Ciò a beneficio della limitazione del consumo di suolo che, per la verità, sta avendo evoluzioni diverse a seconda delle prerogative che hanno avuto le Regioni di

È un passo importante. Non è certamente l'ultimo. Lasciatemi dire perlomeno che dobbiamo agganciare la parte finanziaria.

corposi c'è bisogno assolutamente di un appoggio dal lato finanziario e, pertanto, invito tutti i colleghi ad attivarsi con il mondo finanziario, che fino a questo momento si è dimostrato poco sensibile. Ricordo che negli Stati Uniti ci sono dei prodotti finanziari, che rendono doppia cifra, basati su progetti di efficientamento energetico, mentre da noi i nostri istituti finanziari sono molto più indietro. Ci sarà da lavorare anche per l'incapienza fiscale, che è un altro problema da risolvere. decisamente soddisfatto che dopo tre anni si arrivi a questo risultato che darà decisamente una boccata di ossigeno alla filiera edile e, a cascata, a tutta la filiera economica italiana.

I più recenti dati ISTAT che registrano l'Italia in deflazione, ci confermano quanto sia importante puntare sulle agevolazioni ai consumi, in particolare se queste agevolazioni sono indirizzate alla realizzazione di interventi di efficientamento. ai dati raccolti nel *report* stilato da Cresme e Servizio Studi della Camera sugli effetti delle detrazioni fiscali al 50 per cento per il recupero edilizio e dell'ecobonus 65 per cento per le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 207 miliardi di euro, con una media di 11 miliardi di euro all'anno; Tutte le mozioni intendono prorogare ulteriormente l'ecobonus che, in assenza di estensioni, ritornerebbe dal 2017 all'aliquota prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi che è fissata al 36 per cento e che ha dimostrato di poco efficace rispetto a quella attualmente in vigore. A questo Paese serve una visione politica di lungo respiro, strutturata e che determini cambiamenti reali e definitivi, una vera spinta propulsiva. L'Italia deve crescere, non solo economicamente non possiamo continuare ad andare avanti con *bonus* o politiche a tempo; per raggiungere obiettivi ambiziosi serve una pianificazione. Immaginare il futuro significa essere governanti ispirati, amministrare il presente con *bonus spot* non inseriti a sistema segnala l'incapacità di delineare azioni che vedano il nostro Paese protagonista di un percorso innovativo e di tutela ambientale per le future generazioni.

ad una delle filiere industriali più antiche e, nel contempo, più moderne, efficaci ed efficienti del Paese: quella legata all'edilizia e al suo indotto. Il fatto di voler consolidare questa misura è il segno dell'attenzione del Parlamento e del Governo su una misura decisiva di politica industriale, che quando si vuole si può e si deve fare anche nel nostro Paese

poco, troppo poco, forse si è fatto sul fronte dei consumi. Questa misura è andata in controtendenza. Mentre poco si è fatto sui trasporti (molto si può ancora fare sulla mobilità, sulle città),

di tutte le mozioni. Salutiamo questo voto unanime come un voto importante, che affida al Parlamento e al Governo uno dei temi su cui davvero nei prossimi anni si può consolidare la ripresa di uno sviluppo duraturo per il nostro Paese.*(Applausi

Signor Presidente, ieri il Consiglio d'Europa ha accolto il ricorso della CGIL per il mancato rispetto della legge n. 194 del 1978, questa volta esaminando l'aspetto della discriminazione del personale medico che sceglie di non esprimere l'obiezione di coscienza contribuendo così a garantire un servizio essenziale a tutela del diritto della salute delle donne. Non è la prima volta che il nostro Paese è oggetto di forti critiche perché, non solo non rispetta la legge che si è dato, dopo lunghi anni di battaglie in difesa dell'autodeterminazione della donna, ma viola anche i principi che l'Italia ha fatto propri mediante i numerosi accordi internazionali, tra i quali due patti internazionali nati in seno alle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali e su quelli civili e politici, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000. Diciamo anche che a poco valgono le tiepide giustificazioni del Ministro della salute che, già smentita, ha sostenuto l'utilizzo di dati vecchi, tanto più che la relazione annuale che il Ministero consegna al Parlamento esprime a parole valutazioni non suffragate dai dati inseriti nelle tabelle della relazione stessa. Come si può sostenere che il diritto all'accesso alle tecniche dell'interruzione volontaria di gravidanza sia garantito a fronte di una percentuale di ginecologi obiettori del 70 per cento su scala nazionale,

In generale, numeri a parte, l'Italia non brilla per l'assistenza alla donna, che in certi casi non viene accompagnata con la dovuta attenzione verso un'esperienza traumatica. La sofferenza si avverte anche in alcuni grandi centri urbani. I non obiettori hanno un'età media di sessant'anni; non c'è ricambio proprio perché il servizio viene concepito come negletto, non certo come l'aspirazione di chi, dopo anni di studio e precariato, fa ingresso nel mondo del lavoro. Insomma, l'obiezione di coscienza deve essere disciplinata per evitare che, come accade a Bari, quando l'unico medico non obiettore va in ferie, il servizio sia sospeso, ma anche per evitare che i pochi non obiettori si riducano solo alle interruzioni di gravidanza. Possiamo anche affermare che l'aborto è un male, ma l'aborto clandestino è sicuramente un male peggiore, che espone ad un rischio enorme la donna. L'obiezione di coscienza è accettabile in linea di principio, ma deve essere un'eccezione e non la regola. Ho sollecitato in più occasioni il Ministro, il Governo in generale e il Parlamento su questo tema; ho presentato il disegno di legge n. 923, volto a stabilire una quota minima di personale non obiettore nelle strutture pubbliche; due mozioni, due interrogazioni. Credo sia quanto mai necessario iniziare a parlare seriamente delle azioni da mettere in atto per garantire che la legge n. 194 venga applicata davvero. Non dovevamo forse mettere al centro della nostra sanità il paziente, oppure la nostra è sempre una sanità medico-centrica? Cominciamo a ragionare su questo.

che ha recepito parzialmente il *bail in*, 140.000 risparmiatori tra azionisti e obbligazionisti hanno perso tutto; molti i risparmi di una vita. Solo per gli obbligazionisti subordinati si sta parlando di circa 300 milioni persi. Il Governo non prevede in quel decreto alcun ristoro. Nascono le proteste fuori dall'Aula da parte dei risparmiatori; anche in Parlamento da parte dei Gruppi della Lega Nord. Poi c'è il travaso del decreto-legge nella legge di stabilità. Dopo tante proteste, spunta un fondo di solidarietà di 100 milioni, decisamente insufficiente. In parallelo al fondo di risoluzione, nasce anche la previsione dell'arbitrato: una pessima scelta che introduce discrezionalità perché presuppone comunque l'accertamento di responsabilità in seno a funzionari della banca. Si approva la legge di stabilità; il *premier* Renzi promette all'inizio di gennaio che la partita verrà chiusa entro la fine del primo mese dell'anno. Chiama, nonostante non abbia ancora fatto il san Cantone un'altra volta a fare l'arbitro di questa partita che, ancora una volta, non è una semplice partita, non è una semplice competizione elettorale. Gennaio passa, a marzo circolano voci da parte di esponenti del Governo che dicono che quest'ultimo pensa di ristorare tutto. I risparmiatori truffati si illudono. passa il 31 marzo, che era il novantesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di stabilità, termine ultimo da parte del Governo per emanare il decreto ministeriale che doveva stabilire i criteri dell'arbitrato, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che doveva individuare Siamo al 12 aprile, ben lontani dal 31 marzo, e la legge di stabilità è disattesa: un'altra negligenza da parte del Governo; ancora una promessa vana da parte del Governo e del suo *premier* Renzi. Una nuova promessa disattesa come

e il Monte Senario non ha visto arrivare Renzi a piedi su quella vetta. Quindi questo è un Esecutivo che usa la fretta per varare un decreto nottetempo per tutelare le *lobby* e i banchieri, tra cui anche parenti di autorevoli esponenti del Governo e, a distanza di cinque mesi, non fa nulla per tutelare i risparmiatori. Ci sono quelli di CariFerrara, ci sono quelli della CariChieti, quelli della Banca Marche e soprattutto quelli della Banca Etruria che non sono solo risparmiatori toscani, ma anche di altre Regioni, come ad esempio quelli della cittadina di Pizzoli, dove oltre mille risparmiatori hanno perso i risparmi di una vita. chiusa questa partita? Per questo motivo io ed altri esponenti della Lega Nord abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Padoan con la quale lo sollecitiamo a varare un nuovo provvedimento e, soprattutto, a mettere nero su bianco che il fondo di solidarietà deve essere integrale, pari a 280-300 milioni per prevedere il ristoro integrale di questi risparmiatori truffati. *(Applausi del Presidente, l'INPS il 30 maggio 2014 ha interpellato il Governo, e il Ministro del lavoro in particolare, e ha proposto una soluzione per il pensionamento e il riconoscimento di una maggiorazione di un quinto per tutti i periodi prestati di servizio militare da parte, appunto, degli stessi militari. Non vi è stata alcuna risposta così si va avanti con l'INPS che non riconosce questa anzianità prevista della legge 27 maggio 1977, n. 284, e quindi con le cause successive da parte dei militari, con danno di spese legali e di interessi

alla Presidenza del Senato di intervenire perché questa risposta deve essere data per evitare ulteriori danni e per riconoscere ciò che è previsto dalla legge. Non è un fatto enorme. Possiamo capire che si prenda tempo da anni